pomeridiana di oggi terminerà alle ore 18,30. Informo inoltre, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, che nella seduta di question time di domani alle ore 16, il Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: posizione dell’Italia nell’ambito della strategia di difesa comune europea e dispiegamento del contingente militare italiano in Libia. ordine del giorno: alle ore 9,30 Seguito della discussione dei disegni di legge: Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla

è inteso esclusivamente a favore della produzione indipendente. Crediamo, infatti, che in questo disegno di legge ci si sia già sbilanciati abbastanza in favore della grande distribuzione, delle grandi produzioni e di e di tutte quelle sigle che ben conosciamo e che, come ho già detto, hanno legami finanche parentali con membri del Governo. Cerchiamo, allora, di riequilibrare questo sbilanciamento, perché perché la produzione indipendente, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, costituisce una fetta molto importante dell’industria cinematografica in Italia. «Indipendente» non è sinonimo di «minore»:

quali produzioni e distribuzioni faccia riferimento.

la nuova disciplina del credito d’imposta, il cosiddetto tax credit. Tali articoli individuano, come ho specificato nella relazione iniziale,

dall’intervento di tanti colleghi dell’opposizione, è stato introdotto uno specifico caso per la distribuzione di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana, per potenziare l’offerta cinematografica nelle Regioni italiane dove risiedono le minoranze linguistiche.

per il potenziamento dell’offerta cinematografica italiana ed europea e per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale. Anche questo è un aspetto fortemente innovativo:

c’è l’introduzione del credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore del cinema e dell’audiovisivo che investono per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive: il cosiddetto tax credit esterno. Questo è molto importante, beneficio, la percentuale di credito d’imposta si innalza nel caso in cui ad essere finanziata sia un’opera che ha avuto già accesso ai fondi selettivi,

Signor Presidente, la collega relatrice, senatrice Di Giorgi, ha giustamente sottolineato il passaggio verso il quale ci stiamo dirigendo:

non solo alle produzioni italiane, ma anche alle produzioni estere da realizzare qui in Italia. È il cuore del disegno di legge o comunque ne è una parte sostanziale e voglio intervenire per sottolinearne l’importanza

e bene facciamo ora, anche raccogliendo gli input derivanti dagli emendamenti e dai diversi disegni di legge presentati, ad assegnare a questa materia un corpo più il credito d’imposta per le imprese di produzione, che già esisteva dalla legge del 2007, poi il credito d’imposta per le imprese di distribuzione, anch’esso esistente. In Commissione, in particolare per questo aspetto, è stato introdotto uno specifico caso proprio per le opere prodotte

soprattutto in alcune aree che già si stanno organizzando con le Film commission, dei veri e propri set naturali, con tutto quello che ne può derivare dal punto di vista della creazione di lavoro e di lavoro di qualità. Voglio sottolineare anche la previsione del credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di postproduzione, quindi non si prende in esame solo l’aspetto prettamente artistico, ma anche la possibilità di rafforzare il sistema dell’impresa che di più si occupa degli aspetti tecnici, della parte tecnica di cui la storia del cinema italiano è molto ricca: non abbiamo solo grandi registi e grandi attori, ma anche grandiosi, straordinari direttori della fotografia, sceneggiatori e qui entrano in gioco altre importanti opportunità. Desidero poi sottolineare l’aspetto

si sostiene che non si fa abbastanza per la cultura e che non si investono abbastanza risorse. Ecco, questo disegno di legge, questo importante strumento che andiamo ad approvare, può arrivare complessivamente, già dal 2017, ad impiegare ben 260 milioni di euro rispetto, come si diceva, milioni del 2015. Quindi c’è una lievitazione di opportunità con tutto quello che ne può derivare sia direttamente per le imprese, sia per l’indotto, sia per migliorare la qualità

non solo una valorizzazione di tante imprese, ma soprattutto la creazione di numerosi posti di lavoro.

anche alle imprese di distribuzione di film nella lingua delle minoranze linguistiche. Questo importante strumento anche alle sale cinematografiche e alle imprese di distribuzione situate nelle Regioni dove sono insediate le minoranze linguistiche Per questo motivo, ringraziamo molto la relatrice e anche il ministro Franceschini per la sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche e preannunciamo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

infatti, all’inizio recita: «Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti

confligge linguisticamente con l’introduzione del comma, perché o potenziamo la presenza delle opere o potenziamo la fruizione, ovvero il numero degli spettatori che fruiscono dell’opera. osservazione, a mio avviso, ha fondamento quando decidiamo di prediligere, come parametro, il numero degli spettatori - quindi la quantità della fruizione, un meccanismo legato alla bigliettazione - piuttosto che un parametro di tipo qualitativo, cioè la qualità culturale

di prendere in considerazione l’estensione di questa misura anche a questo tipo di società, fondamentali per la produzione di un’opera audiovisiva e cinematografica.

ma semplicemente perché siamo, lo ribadisco, in un testo normativo e quindi «produzione» ci sembrava e ci sembra un termine comprensivo di tutte le fasi fino alla

Santangelo, non posso decidere da solo, mi consulterò con il Presidente del Senato. Ora verifichiamo il sostegno per questo caso, poi sulla legislatura approfondiremo.

L’industria cinematografica (e non solo) subisce costantemente grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico. In pochi anni siamo passati da una vecchia tecnologia (eccellente, per carità) che che funzionava analogicamente a pellicola, al digitale. Ora, questi macchinari costano decine se non centinaia di migliaia di euro, quindi nessuno si

ma non vedremo mai un film, né potremo girarlo, né potremo proiettarlo. Ora, visto che queste tecnologie subiscono un avanzamento molto rapido (siamo passati dalla vecchia immagine analogica standard defini_tion, quella che vedevamo un po’ sgranata, al 4K,

introdurre questo parametro senza un correttivo significa che, automaticamente, i sostegni da parte dello Stato finiranno a quei film che potranno godere di una rete distributiva più potente rispetto ad altri film, magari di qualità anche superiore, ai cosiddetti blockbuster. Non abbiamo nulla contro i blockbuster, ma nel corso delle audizioni svolte durante l’esame di questo provvedimento spesso è stato portato come esempio come esempio un fenomeno eclatante per quanto riguarda il mondo del cinema, ovvero il grande successo che ha avuto il film di Checco Zalone all’inizio di quest’anno. successo è stato sicuramente dovuto alla qualità del film e alle qualità di Checco Zalone, ma anche al fatto che il film è stato distribuito in migliaia di sale cinematografiche negli stessi giorni, a discapito della programmazione di altri film, probabilmente considerati

sicuri davvero di dare l’opportunità a tutti i film, anche ai non blockbuster, di ottenere finanziamenti in base alla qualità dell’opera.

seppur condivisibile su tutto il fronte, non opportuna in questo caso.

parla del rapporto tra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione. Se la relatrice riesce a trovarmi nel testo dell’articolo 22 le modifiche che possono soddisfare la preoccupazione rappresentata da questo emendamento e i correttivi che esso vuole introdurre, ne sarei ben felice sarei disposta a ritirarlo. Siccome sono convintissima che non sia così, invito i colleghi a votare favorevolmente perché su questo si gioca il futuro di una parte del nostro cinema, del cinema culturale e di qualità.

quote di riparto siano assegnate ai settori relativi all’ideazione e alla stesura, alla produzione e alla postproduzione.

che venisse considerato il complesso della produzione.

l’emendamento 24.10 mira ad ampliare i requisiti per le opere audiovisive che possono accedere ai contributi selettivi e in particolare per quelle opere audiovisive che hanno come intento la promozione di temi di rilevanza sociale quali ad esempio il bullismo, il cyberbullismo, il femminicidio, l’educazione

permetto anche di illustrare con forza questo emendamento nella speranza che il plafond si possa ampliare. Ma l’emendamento sul quale mi voglio concentrare

del comma 4, quella di rendere strutturale l’intervento previsto da questo provvedimento, eliminando il deferimento a una decretazione ministeriale, ma facendo diventare queste misure strutturali. Come sappiamo, quando si opera nel campo cinematografico e si fanno investimenti soprattutto nella produzione di un film, ma anche nella distribuzione nelle sue varie fasi, è importante sapere che che si potrà contare su incentivi fiscali o comunque su misure tese ad aumentare il sostegno al comparto. Il fatto di rendere strutturali queste misure chiaramente aumenta il grado di certezza e quindi anche il grado di partecipazione e di investimento nelle opere audiovisive e cinematografiche. Senza questa certezza si verificano quei fenomeni, ai quali siamo abituati, di scarsa propensione all’investimento proprio dovuto ad un’incertezza dei sostegni ai quali si potrà accedere. Tradotto in pochi termini, se so che potrò usufruire di determinati sostegni finanziari allora sarò maggiormente incentivata ad investire; se invece corro il rischio di ritrovarmi priva di questi sostegni per un’intervenuta modifica ai decreti ministeriali, allora è chiaro che questa propensione all’investimento cala.

dell’articolo già si richiamano le competenze riconosciute a livello internazionale; inoltre, queste due paroline «chiara fama» in altri contesti hanno aperto la porta a personaggi che poi tanto di chiara fama non erano. Siccome le leggi sono interpretabili e non vogliamo che si corra questo rischio, ci asterremo - ripeto - su questo emendamento, pur concordando sul fatto che gli esperti debbano avere una comprovata e riconosciuta competenza, come peraltro

perlomeno, di riconoscere le qualità creativo-professionali, altrimenti rischiamo di non valorizzare

anche a opere cinematografiche che hanno una possibilità di divulgazione a livello didattico nelle scuole, quindi di incentivare quello che anche il testo nel suo complesso vorrebbe ottenere, cioè che le produzioni cinematografiche culturali e di qualità vengano poi diffuse soprattutto tra i giovani,

automatici, si definiscono i requisiti minimi che devono possedere le imprese, i criteri di assegnazione dei contributi, il termine massimo entro cui l’importo può essere utilizzato e i casi di decadenza ovvero di revoca. Quanto ai contributi selettivi,

dire abbiamo pensato di inserire all’interno di questi contributi selettivi - che possono essere anche amplificati da un’importante relazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulle modalità

cioè di questo pilastro previdenziale. Poi si è deciso, fortunatamente per i nostri padri, che non bisognava assolutamente dare questo sistema in mano ai privati. Gli anni passano, però, e si è creato un nuovo sistema, il sistema previdenziale integrativo (non si è toccata, fortunatamente, la base),

è totalmente in mano al sistema privatistico ed è volontario.

Questa è una cosa pericolosissima! Stanno facendo entrare banche e assicurazioni nel nostro sistema previdenziale pubblico. Signora

sull’utilizzo del deposito che dovremo costruire per i rifiuti radioattivi. Parliamo ancora una volta di questa eredità di una sciagurata politica energetica del passato che ci perseguiterà (e confermo il verbo «perseguitare») per i prossimi 200.000 anni. Non è una cifra a caso, sono dati scientifici: i rifiuti radioattivi impiegano infatti 200.000 anni per perdere la loro mortale pericolosità.

ma non si capisce esattamente né in quale quantità né come sia stato gestito. In particolare, ho chiesto quale sia l’organo terzo, e quindi estraneo all’amministrazione della Difesa, che vigila sulla corretta gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle nostre forze militari. Pertanto, da una parte, abbiamo una situazione per la quale lo smantellamento delle centrali nucleari e la costruzione del deposito di rifiuti procede con estrema lentezza (anzi manca ancora il piano nazionale quindi siamo proprio privi

un argomento probabilmente divisivo e quindi viene rimandato: facciamo finta che il Parlamento non lavori quando invece il Parlamento è messo sotto scacco da un Governo che utilizza queste tecniche per non farlo lavorare. Lo dico

Queste sono veramente misere strategie di comunicazione che non fanno lavorare il Parlamento e non permettono un miglioramento della vita dei cittadini.

da parte del Ministro e da parte di quel programma Centostazioni (e mi rivolgo anche al ministro Franceschini, che è di Ferrara, vicino a Rovigo), la stazione di Rovigo a tutt’oggi ha tutte le sue barriere architettoniche.

persone portatrici di handicap, delle persone disabili, delle persone con difficoltà di deambulazione, delle persone ipovedenti e non vedenti, delle persone anziane, delle persone con bagagli (ne possiamo aggiungere finché vogliamo). Io reputo che sia una cosa vergognosa che nella stazione di

se il Regolamento è un optional perché evidentemente per questo Governo lo è, non può essere un optional abbattere le barriere architettoniche, ma una necessità. Sollecito

sia al Ministero dello sviluppo economico il reinserimento della mia città, la città di Sulmona in Provincia dell’Aquila, nei poli di attrazione. Per motivi a noi sconosciuti la mia città era nei poli di attrazione, ma

Chiedevo appunto che la mia città venisse reinserita, avendo tutte le caratteristiche per poter essere oggi un polo di attrazione.

e molto attuale, concernente un episodio francamente sconcertante. Nella città di Prato, un gruppo di giovani di Forza Italia ha

Sicuramente è un contenuto opinabile, ma per l’appunto siamo nella libertà di espressione. Questo manifesto è stato tagliato materialmente da

reato esprimere critiche, peraltro contenutissime, nei confronti del Presidente del Consiglio. Siccome il Presidente del Consiglio era a Prato per fare propaganda per il sì al referendum, mi pare che questo sia doppiamente grave, in quanto comporta la violazione della libertà di espressione e la

di questo manifesto e, per di più, il fatto che ne abbiano lasciato un pezzo appeso dimostra che era affisso legalmente: non vi era alcun problema di autorizzazione, di bolli, di timbri o di chissà che.

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento al Ministro della difesa sui seguenti argomenti: - posizione dell'Italia nell'ambito della strategia di difesa comune europea - dispiegamento del contingente militare italiano in Libia La seduta è tolta